che parafrasava il motto voluto dai nazisti all'ingresso del *lager* di Auschwitz e suggeriva un'analogia tra le azioni delle SS e le scelte del Governo israeliano.

televisione a prendere posizione a nome anche, a mio giudizio, di buona parte di questa maggioranza. Noi non abbiamo mai sentito scuse dal direttore Sansonetti, che si è limitato, il 16 maggio, a sostenere che la vignetta era molto dura e scioccante, ma certamente non era antisemita. Non sono arrivate parole di rimprovero da parte del segretario di partito; a questo punto, è evidente che si pone il problema di un chiarimento da parte del Governo e della maggioranza

Aggiungo un elemento, signor Presidente, che è più attuale e su cui il Sottosegretario non si sottrarrà ad un confronto, al di là delle carte scritte, cioè sulle manifestazioni.

ben chiari, come la richiesta degli organizzatori di azzerare i trattati di cooperazione con Israele. L'unico partecipante che ha avuto il coraggio di prendere una posizione di equidistanza

non si considerano però i missili che, quotidianamente. colpiscono Israele; non si considera il caso di Gaza. è un'occasione sprecata per la causa palestinese. Gaza è stata restituita alla causa palestinese credo con grande sacrificio da parte di Israele. Ricordo i pianti, ricordo l'esercito israeliano che strappava da quella terra i propri fratelli per una scommessa, per un'ipoteca sulla pace. Ebbene, da Gaza

Il Governo italiano ritiene che l'episodio evocato nell'interpellanza non possa essere inteso in alcun modo come "l'atto d'avvio di un nuovo atteggiamento nei confronti della comunità ebraica di posizione antiisraeliana per quel che riguarda la situazione in Medio Oriente". La questione israelo-palestinese non si presta a semplicistiche posizioni «pro» o «anti» qualcuno. L'Italia ha storici e profondi rapporti di amicizia e solidarietà con Israele e con il popolo palestinese. E' un patrimonio di credibilità, di serietà e di impegno che questo Governo intende coltivare e valorizzare, non certo disperdere. La vignetta in questione intendeva presumibilmente denunciare, in forma paradossale e grottesca, l'occupazione israeliana, la barriera di sicurezza, le pressioni economiche nell'attuale congiuntura palestinese su una popolazione già povera e quindi il rischio di una catastrofe umanitaria nei Territori palestinesi che, in sede europea, siamo impegnati a scongiurare. Purtroppo, con il richiamo ad Auschwitz, l'autore è andato deplorevolmente oltre il bersaglio ed è più che comprensibile che la comunità ebraica ne sia rimasta sensibilmente offesa. Il parallelo fra il campo di sterminio di Auschwitz e l'occupazione israeliana in Cisgiordania è certamente offensivo e grottesco, ma ovviamente esso impegna solo quel vignettista e il giornale che ha ritenuto di pubblicare la vignetta. L'attuale Governo, come, del resto, quelli che lo hanno preceduto, ha sposato la causa di una pace giusta e negoziata, che ponga fine al tragico conflitto tra i due popoli e avvii una convivenza potenzialmente in grado di condividere progresso e benessere. Oggi questa soluzione si incarna nella prospettiva bi-statuale, contenuta nella Roadmap adottata da Stati Uniti, Russia, Unione Europea e Nazioni Unite: due Stati indipendenti e sovrani, Israele e Palestina, che si riconoscano reciprocamente, che possano convivere fianco a fianco in sicurezza, armonia e collaborazione. Il Governo si muove in quest'ottica - credo che ciò sia stato evidente anche nelle valutazioni che ha espresso in occasione delle recenti manifestazioni, come lei stesso ricordava - e farà quanto è in suo potere, razionalmente ed in seno all'Unione Europea, perché si avanzi verso questo traguardo.

Lavignetta appartiene sicuramente al giornalista e al direttore; ricordo però che questo non è un giornale

è un problema politico come dice giustamente Furio Colombo, che prosegue: «una vignetta è spesso il più folgorante degli editoriali. Assisto con sgomento al fatto che la sinistra, quella parte che ha offerto vite,» non solo di sinistra, aggiungo io - «anni di carcere e la più dura delle resistenze per combattere il nazismo, possa compiere oggi questo curioso atto di incoscienza». aggiunge che la questione non riguarda solo Rifondazione, bensì «tutti quelli che si sentono parte del centro-sinistra (...). È come l'umidità di casa: se c'è una macchia in un angolo tutta la struttura deve essere rivista». non drammatico, ma sicuramente reale, di un antisemitismo che sta prendendo piede in Europa e anche nel nostro Paese: il 10 luglio scorso alcuni personaggi hanno imbrattato i muri del quartiere ebraico di Roma con svastiche naziste,

al tavolo della consulta islamica. L'Ucoii ha marciato ad Assisi per la pace con le foto di Nasrallah, *leader* di Hezbollah. Il problema è quindi politico e va affrontato in modo complessivo. Lo dico sommessamente, ma con molta convinzione. Signora Sottosegretario, quando lei parla di «pace giusta e negoziata», pensiamo forse - lo pensa il suo ministro D'Alema - che sia un problema di terra e che concedendo o togliendo, in questo fazzoletto di terra - ahinoi - non più grande del Lazio, un metro o un altro metro, si possa arrivare, con uno sforzo, alla pace. Leiha parlato di riconoscimento: «due Stati che si riconoscono». L'ho già letto, ma lo voglio rileggere, perché credo che forse farebbe bene a tutti

e i musulmani non li uccideranno e fino a quando gli ebrei si nasconderanno dietro una pietra o un albero, e la pietra e l'albero diranno: "O musulmano, o servo di Allah, c'è un ebreo nascosto dietro di me, vieni e uccidilo"...». Ecco, questo è lo Statuto del movimento di Hamas. possiamo pensare: due Stati, un'uguale distanza tra un movimento che prevede di uccidere tutti gli ebrei e che non avrà realizzato il suo Statuto finché non sono tutti morti e uno Stato democratico,

una manifestazione-corteo dei reduci della Repubblica di Salò insieme ad alcune centinaia di manifestanti. Questa manifestazione, che è altamente offensiva per i cittadini e le cittadine scledensi, che si sono distinti in particolare modo nella lotta antifascista, prende a pretesto il ricordo dell'eccidio avvenuto, per mano di un gruppo autonomo di partigiani non legati a catene di comando, nelle carceri di Schio nel luglio del un triste episodio che costituisce ancora una ferita profonda nella coscienza civile e nella memoria di questa città. Con l'alibi della commemorazione, però, ogni anno il Sacrario militare e l'intera città di Schio diventano teatro di una vera e propria gazzarra di stampo nazifascista che offende insieme alla città anche i familiari e gli eredi delle vittime, che non si sentono rappresentati da quei figuri e si dissociano pubblicamente da tale strumentalizzazione che offende poi, in particolare modo, anche la memoria dei tanti partigiani che sono sepolti in quel Sacrario. Il ricordo di quell'eccidio esecrabile, infatti, è diventato la scusa per una strumentalizzazione politica durante la quale si inneggia al nazifascista con *slogan*, gesti e simboli inequivocabili, dal saluto romano al grido «boia chi molla», dalle bandiere della Repubblica sociale italiana, all'accusa di assassini rivolta alla generalità dei cittadini di Schio. Tutto quello che sto dicendo è ampiamente documentato negli anni da foto apparse sulla stampa locale e che sono in possesso anche delle forze dell'ordine e che, a mio avviso, sarebbero più che sufficienti per impedire una manifestazione che evidentemente qualche problema di ordine pubblico lo crea. Questa manifestazione, invisa ai cittadini, è avversata da tutte le forze democratiche, tanto che fin dal 2005 il Sindaco, le associazioni partigiane e il Comitato dei familiari delle vittime hanno firmato un documento comune dichiarano di riconoscersi nei valori fondanti della Repubblica italiana e della Resistenza, condannano l'eccidio di Schio ad opera dei partigiani, promuovono la memoria dei 54 trucidati e invocano la concordia civica dissociandosi da ogni offensiva manifestazione che strumentalizza i morti di quell'eccidio. Nel luglio scorso, il Governo e le diverse autorità preposte hanno ricevuto diverse sollecitazioni, a partire da quelle del Sindaco, rivolte ad evitare, ancora una volta, lo svolgimento di questa manifestazione pubblica. Anch'io, insieme alle altre parlamentari venete del centro-sinistra, con una lettera, il 23 maggio, avevo rivolto un appello al Ministro dell'interno affinché impedisse che venisse nuovamente tradito per la quinta volta di seguito da una manifestazione e un corteo palesemente pretestuosi ed inneggianti al nazismo e al fascismo lo spirito di quel solenne documento firmato dai familiari degli uccisi, dalle associazioni partigiane e dal Sindaco. In effetti, dopo numerosi e reiterati incontri con il prefetto e il questore, nel luglio scorso, non è stata autorizzata alcuna manifestazione, ma tale divieto è stato bellamente aggirato con la richiesta al al Comitato per l'onore dei caduti in guerra, che gestisce i Sacrari militari, dell'uso del Sacrario per il pretestuoso svolgimento di una pseudomanifestazione religiosa. Dico «pseudomanifestazione» senza ovviamente alcuno intento polemico e di non rispetto, ma perché il sacerdote che l'ha guidata è un ex-sacerdote sospeso *a divinis*, quindi di manifestazione religiosa non possiamo parlare. Devo dire, poi, che la richiesta di uso del Sacrario è stata presentata dal referente locale di un'associazione che si nomina «Continuità ideale con la Repubblica sociale italiana». Penso che solo la firma di quel documento sia un reato e che una simile sigla non possa essere tollerata nella Repubblica italiana. In considerazione dei precedenti, il 5 luglio avevo presentato un'interpellanza per chiedere, appunto, che venisse negato anche l'uso del Sacrario che avrebbe potuto consentire, come poi in effetti è avvenuto, è avvenuto, una manifestazione con corteo non autorizzato. Ma, evidentemente, il nuovo Governo era da troppo poco costituito (aveva ottenuto da pochissimo la fiducia) e non c'è stato il tempo materiale di intervenire. Come era prevedibile, i partecipanti hanno dato vita a un corteo di stampo nazi-fascista, hanno diffuso *slogan* inneggianti alla violenza e all'intolleranza e addirittura - io stessa sono in possesso di fotografie che potrei fornire in qualsiasi momento - hanno issato sul pennone del Sacrario militare, accanto al tricolore italiano, il famigerato e triste vessillo della Repubblica sociale. Le forze dell'ordine, che pure sono prontamente intervenute, al comando del questore di Vicenza, per evitare la manifestazione non autorizzata, non hanno però potuto evitare un corteo, aperto dall'europarlamentare Alessandra Mussolini e da noti esponenti di Alternativa sociale provenienti da tutta Italia, che dal Sacrario si è portato alle ex carceri mandamentali, luogo dell'eccidio. In testa a questi manifestanti, come gli altri anni, c'era questo sedicente padre Giulio Tam, sacerdote sospeso *a* *divinis*, che, giunto alle carceri, ha letto l'appello delle 54 vittime della strage del 7 luglio 1945. A ogni nome devo dire che per ultimo è stato fatto quello di Benito Mussolini, che alla data del 7 luglio 1945 era comunque già morto - è seguito il grido «Presente», condito dal saluto romano. Poi, la manifestazione non autorizzata è ritornata al cimitero ossario per una messa di suffragio con rito preconciliare. Anche quest'anno Schio è stata completamente blindata e sorvegliata dal basso e dal cielo da oltre 500 carabinieri, poliziotti, finanzieri e vigili urbani e ha dovuto assistere alla macabra ripetizione di ogni peggior ciarpame fascista, all'ostentazione di tristi simboli (c'era una selva di gagliardetti e bandiere), a provocazioni e a risse. Non approvo e non giustifico alcun gesto e comportamento violento, ma, certo, non è possibile non riconoscere le provocazioni costruite a tavolino da chi, in divisa nera e ostentando una vistosa croce celtica al collo, ha cercato di far passare gli altri come violenti.

sua denuncia è stata smentita, anche per quanto riguarda questo episodio marginale, dalle registrazioni che dimostrano come le forze dell'ordine abbiano impiegato esattamente tre secondi a intervenire. stata un'altra aggressione vicino all'ossario; è stato aggredito un ragazzo di passaggio, il figlio ventenne dell'assessora ai servizi sociali, reo, a quanto pare, di indossare una *t-shirt* di Emergency. Rifondazione comunista, i Comunisti italiani, i Verdi, l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, la CGIL, la CISL, la UIL, i CUB e varie sigle dell'associazionismo democratico antifascista, hanno organizzato per quella stessa mattina una contromanifestazione con comizi e concerto, cui hanno partecipato oltre un migliaio di persone che hanno scelto di non lasciare la città in mano ai nostalgici del fascismo, che si sono presentati in alcune centinaia. Assenti erano i cittadini di Schio, che hanno così lanciato un messaggio chiaro: si sono chiusi in casa perché quella città non sopporta questa manifestazione e la strumentalizzazione di un dolore ancora vivo e presente. L'eccidio è una ferita che si sta rimarginando, ma il processo non viene certo aiutato se ogni anno continua a ripetersi una manifestazione tesa a riportare indietro le lancette della storia a un momento definitivamente cancellato dalla Resistenza e dalla Costituzione. Chiedo quindi al Governo, intanto una valutazione sui fatti che anche quest'anno, purtroppo, abbiamo dovuto vedere davanti ai nostri occhi e, poi, di impegnarsi fin da ora, proprio alla luce di quanto in questi cinque anni è avvenuto, per adottare le misure più opportune e la dovuta concertazione tra i Ministeri (non vorremmo, cioè, ancora una volta, che il Ministero dell'interno vietasse ciò che il Ministero della difesa concede) al fine di evitare, del prossimo anno, una manifestazione e un corteo che, con il pretesto anche di una manifestazione religiosa, si trasformano invece in propaganda becera dell'ideologia nazifascista e offendono i sentimenti democratici di tutti i cittadini.

il movimento «Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana» ha annualmente organizzato a Schio una manifestazione in ricordo dei fatti avvenuti tra il 6 e il 7 luglio 1945, quando 54 persone, parte delle quali aderenti alla Repubblica sociale, furono uccise all'interno del carcere di quel centro, ora adibito a biblioteca comunale. La manifestazione si articolava in due fasi: un momento religioso, con una messa al Sacrario militare di Schio, ed un momento più pubblico, con un corteo per le vie cittadine, che negli anni scorsi ha però costituito occasione per momenti di tensione e gesti di intolleranza politica. Anche quest'anno, nelle intenzioni dei promotori, la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi con le stesse modalità, ed in tal senso il 3 luglio era stato presentato formale preavviso al questore, ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Già il 6 giugno precedente, peraltro, analogo avviso, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, era stato presentato per una contromanifestazione promossa dalla sezione locale del Partito della Rifondazione Comunista. Per evitare possibili contrapposizioni e turbative all'ordine pubblico, e tenuto conto anche dei precedenti degli anni scorsi, Questore di Vicenza ha quindi deciso di vietare entrambi i cortei, alla luce anche delle valutazioni espresse dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 6 luglio. Il divieto di sfilare per le vie del centro non riguardava la funzione al Sacrario, anche per non comprimere la libertà costituzionalmente garantita di culto e di espressione religiosa. Ciò nonostante, la mattina del 9 luglio, nelle adiacenze del Sacrario militare, i partecipanti alla messa hanno dato luogo a manifestazioni esteriori inneggianti al fascismo, cercando di dirigersi ugualmente verso il centro cittadino. Le forze dell'ordine, create le necessarie condizioni di sicurezza, sono subito intervenute per indurre i manifestanti a sciogliere il corteo e a fare rientro nel Sacrario, avviando i necessari accertamenti volti ad individuare e segnalare all'autorità giudiziaria i responsabili dei reati commessi di violenza a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata. Le autorità giudiziarie civile e militare sono state, inoltre, informate in merito all'esposizione presso il Sacrario militare di un vessillo della Repubblica sociale italiana e di alcune locandine che riportavano l'immagine del sindaco di Schio e scritte ingiuriose. Aquesto riguardo, dalle informazioni assunte si è appreso che il piccolo vessillo era stato issato su un pennone laterale del Sacrario, sin dalle primissime ore del mattino, da alcuni esponenti del sodalizio promotore dell'iniziativa. L'ufficiale responsabile del Sacrario aveva subito richiesto all'Unione Combattenti della Repubblica sociale italiana la spontanea rimozione sia del vessillo che delle locandine, ma senza ottenere alcun risultato. Come ho detto, anche questa azione è stata sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Si consideri che le autorità locali ritengono che l'aver soprasseduto alla rimozione forzata del vessillo abbia, con ogni probabilità, contribuito in modo determinante ad evitare più gravi turbative dell'ordine pubblico. Preciso, infatti, che nell'occasione non si sono avuti ferimenti o lesioni né tra i manifestanti, né tra le forze dell'ordine, a conferma della prudenza, professionalità e competenza alle quali è stata improntata, anche in questa occasione, la gestione dell'ordine pubblico.

per l'approfondita analisi di quanto successo. Non posso, però, dichiararmi sino in fondo soddisfatta, visto che non mi viene detto che cosa avverrà il 7 luglio del prossimo anno. E' un pochino presto ed abbiamo il tempo per ragionarci, ma mi sembra di vedere, anche dalla risposta che lei mi ha dato, che gli elementi per valutare un pericolo imminente da questa manifestazione ci siano. Mi sembra poi che utilizzare la parola «prudenza» nel non togliere la bandiera della Repubblica sociale italiana che, a me sembra, ai sensi della nostra Costituzione, sia vietata in Italia, così come la ricostituzione del Partito fascista e ammennicoli vari, sia un po' troppo prudente, nel senso che credo che dovremmo avere una posizione molto più ferma e più precisa nel vietare queste manifestazioni. Ricordo poi che, proprio nel nascondersi dietro ad una manifestazione di tipo religioso che - ripeto - per quanto sia poco esperta della materia, non possiamo definire tale se officiata da un sacerdote sospeso *a divinis*, non trova alcuna giustificazione dal momento che i parenti stessi delle vittime si sono sempre rifiutati di partecipare a questa manifestazione, che dovrebbe essere in memoria dei loro congiunti, ed hanno anche quest'anno fatto

ingiustamente uccise. Dico ingiustamente perché qualsiasi morte venga posta, senza un regolare processo, anche in tempo di guerra, è evidentemente fuori da ogni regola e da ogni accettazione da parte di chi intende portare avanti una convivenza di civiltà. - ripeto - non ha nulla a che vedere con la memoria dei morti, ma ha a che vedere solo con una occasione di manifestare l'adesione ai simboli, alle ideologie del disciolto, per fortuna, Partito fascista. fascista. Mi auguro e mi impegno - non so se è una promessa o una minaccia - con il Governo a non far trascorrere un attimo, da oggi al 7 luglio, perché questa manifestazione non tenga - ovviamente insieme alla Giunta, al Sindaco e alle forze politiche democratiche di Schio - perché credo che davvero si tratti di un'ingiustizia che la città ed i cittadini di Schio stanno subendo, tanto che ormai, negli ultimi anni, essi stessi si chiudono in casa ed osservano allibiti, disgustati e direi anche un po' impauriti questa gazzarra inaccettabile nelle loro vie. Ricordo che Schio è medaglia d'argento al valore militare per le gesta compiute durante la Resistenza e, come tutto il resto del nostro Paese, non si merita certo manifestazioni di questo tipo.

per l'interno*. In data 14 aprile 2003, a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione apertura Sale cinematografìche, la Direzione generale per il cinema ha rilasciato autorizzazione alla Tradital S.p.A. per l'apertura della multisala Camerlata 2000 in Como. L'autorizzazione è stata rilasciata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 391 del 1998, sul presupposto che la multisala era inserita nell'ambito di un centro commerciale. Nel mese di settembre 2005 sono state presentate varie istanze, da parte della Cinestar immobiliare s.r.l e dell'Astoria s.a.s, con le quali veniva chiesto l'annullamento del decreto di autorizzazione della multisala Camerlata 2000, in quanto non inserita nell'ambito di un centro commerciale. La Direzione generale per il cinema, dopo aver acquisito informazioni presso le competenti autorità locali, ha ritenuto opportuno predisporre una visita ispettiva. L'ispettore incaricato, a conclusione di indagini accurate, ha affermato che sull'area in questione non era stata rilasciata alcuna autorizzazione avente ad oggetto l'apertura di un centro commerciale. II Ministero per i beni e le attività culturali ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla sussistenza, nella fattispecie, del presupposto dell'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento o alla revoca dell'originario L'Avvocatura generale dello Stato non ha tuttavia ravvisato nell'attività della direzione generale per il cinema violazioni di legge, né altri profili di illegittimità tali da giustificare l'adozione di un atto di annullamento in via di autotutela. L'operato dell'Amministrazione nella fase procedimentale che ha preceduto l'emanazione dell'atto di autorizzazione è infatti apparso all'Avvocatura generale dello Stato del tutto esente da censure. La circostanza del mancato inserimento della multisala nell'ambito di un centro polifunzionale qualificato come centro commerciale, appurata in tempi largamente posteriori alla data di emissione del provvedimento autorizzatorio, potrebbe tuttavia rilevare - a giudizio dell'Avvocatura generale - ai fini di una ipotetica revoca dei provvedimento stesso, qualora si dovesse ravvisare nella fattispecie in esame l'esigenza di una nuova valutazione dell'interesse pubblico a causa del mutamento della situazione di fatto. Tuttavia, l'Avvocatura generale dello Stato ha puntualizzato che l'interesse pubblico attuale oggetto di tale nuova valutazione - che potrebbe portare alla revoca del provvedimento autorizzatorio - è, nella specie, riconducibile anche alla sfera di interessi di competenza delle amministrazioni locali. La Direzione generale per il cinema ha quindi contattato il Comune di Como e la Regione Lombardia al fine di valutare la sussistenza o meno di un interesse pubblico attuale alla revoca del provvedimento amministrativo con il quale è stata autorizzata l'apertura della multisala Camerlata 2000. Ad oggi non è ancora pervenuto riscontro da parte delle amministrazioni locali.. Il Comune di Como ha tuttavia comunicato che il consiglio comunale, nella seduta dell'11 settembre 2006, ha disposto di approvare, ai sensi delle leggi regionali n. 23 del 1990 e n. 12 del 2005, modifiche al piano integrato di recupero edilizio ed urbanistico «ex Trevitex», con contestuale adozione della variante urbanistica proposta dalla società CEDI srl, per l'ambito ubicato in Como, Via Paoli n. 6. La predetta approvazione costituisce la prima tappa dell'*iter* necessario ai riconoscimento della natura di centro commerciale (dal punto di vista urbanistico) del complesso nel cui ambito è inserita la multisala Camerlata 2000 Europlex 9. Tale *iter* proseguirà attraverso successive fasi, fino alla eventuale definitiva approvazione regionale del piano. Pertanto, tenuto conto che la procedura di cui sopra è tuttora in corso, si ritiene indispensabile attendere l'esito della procedura in atto presso il Comune di Como prima di valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti in merito.

Lei sa che questa è una storia cominciata alla Camera dei deputati, dove era proprio il suo omologo ai Beni culturali a rispondermi e lo faceva sempre, come ha fatto anche lei, con dovizia di particolari, a volte anche molto duramente e rigorosamente.

il problema è il gioco delle scatole cinesi, che lei ha ricordato, in cui le società compaiono e scompaiono quasi fossero oggetto di giochi di prestigio. Gli ispettori del Ministero hanno rilevato l'inesistenza di un centro commerciale in quella struttura e quindi l'assenza dei presupposti stabiliti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un cinema multisala, ma lì il cinema multisala opera da tempo. struttura non può esserci un centro commerciale perché il Consiglio comunale di Como, il 30 ottobre del 1997, escluse specificamente la destinazione di quell'area a centro commerciale.

Poi, però, il Consiglio provinciale - e qui vi sono omissioni nella risposta del Ministero - ha votato una mozione che evidenzia come il centro commerciale, con annessi e connessi, non sia minimamente previsto nel PTCP, L'illegittimità che si è consumata è totale, evidente, direi beffarda nei confronti del Ministero e dell'Amministrazione, che è stata presa in giro da un Comune i cui uffici hanno espresso opinioni discordanti in più di un'occasione. Le sue risposte sono precise per un verso ed evasive per l'altro e mettono una pietra sulla legalità ed il rispetto delle regole: questo francamente mi spiace.

L'atto oggi in discussione prende spunto dall'incidente che il 22 maggio scorso ha visto coinvolti due F16 dell'Aeronautica militare italiana, per affrontare, in generale, il tema della presenza militare in Sardegna e dei vincoli territoriali derivanti dai poligoni militari e dalle aree utilizzate per le esercitazioni militari e, nel contempo, ipotizzare disagi di ordine economico, industriale e turistico per le comunità locali più direttamente coinvolte dalle attività addestrative delle Forze armate. In primo luogo, sull'incidente il Governo ha già chiarito in Parlamento, nella seduta della Camera dei deputati del 23 maggio scorso, che i due velivoli da caccia monoposto F16 sono precipitati a causa di una collisione in volo a Largo di Capo Carbonara, durante una missione di addestramento nell'ambito dell'esercitazione multinazionale «*Spring Flag*». Nel ribadire che l'incidente non ha causato danno alcuno a persone o cose, si rimarca che le misure di sicurezza che si adottano per lo svolgimento delle attività addestrative tendono proprio ad evitare possibili danni collaterali. A questo punto, prima di passare ad esaminare in sequenza le singole questioni poste dai senatori interroganti, è opportuno richiamare in sintesi gli aspetti più salienti relativi alla presenza militare sul territorio nazionale, illustrati dal Ministro della difesa nel corso della specifica audizione del 25 ottobre scorso presso la Commissione difesa della Camera dei deputati. In tale sede è stata sottolineata la ferma intenzione del Governo di procedere ad un'attenta valutazione della presenza militare nelle nostre Regioni - ivi compresa naturalmente la Sardegna nell'ottica di una più equa distribuzione degli oneri da essa derivanti, fatta salva, naturalmente, la compatibilità di ubicazione delle strutture in rapporto ai programmi di difesa in linea con l'attuale scenario strategico - e nel rispetto delle legittime aspirazioni di sviluppo civile ed economico delle popolazioni interessate. In tale prospettiva la Difesa ha già avviato un particolareggiato censimento di tutte le infrastrutture e del loro attuale utilizzo, nonché delle servitù ad esse eventualmente associate così da poter acquisire gli elementi indispensabili per modificare quei casi in cui il peso delle attività militari sia eccessivamente concentrato su alcuni territori. In ogni caso, si intende rivedere l'intera materia in una nuova conferenza nazionale che coinvolgerà naturalmente l'Amministrazione della difesa, l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali per una migliore e reciproca comprensione ed una ottimizzazione delle attività. Quanto, in particolare, alla regione Sardegna, l'oggettiva situazione di disagio del territorio sardo è stata pubblicamente riconosciuta dal Governo ed è oggetto di confronto operativo sulla base di una piattaforma concordata con la Regione autonoma della Sardegna. Per quanto concerne le servitù militari propriamente dette - territori estranei al demanio militare ma gravati da limitazioni alla libera fruizione - l'orientamento della difesa è di eliminare quelle che non risulteranno più necessarie, ovviamente, non appena completato questo censimento. Saranno anche vagliati con attenzione i criteri di compensazione previsti dalla vigente normativa per un eventuale aggiornamento degli indennizzi ai privati e dei contributi agli enti locali, compresi gli aspetti procedurali che appaiono ancora molto complessi. A tal fine, ha già iniziato ad operare il gruppo di lavoro Difesa-Regione Sardegna, istituito per affrontare le problematiche di armonizzazione tra le esigenze della Regione e quelle della difesa in materia di servitù militari e di utilizzo delle aree demaniali, definendo congiuntamente gli obiettivi finali, i criteri di soluzione e le tempistiche ad essa associate. In particolare, per il poligono del Salto di Quirra si è deciso di procedere ad ulteriori verifiche, su base concordata, in merito allo stato ambientale dello stesso e delle zone limitrofe. La difesa ha ad essi manifestato la propria disponibilità ad approfondire le possibilità di bonifica delle aree marine prospicenti il poligono di Capo Teulada dove ad oggi, tuttavia, non è risultato che sussista alcuna situazione pregiudizievole per l'ecosistema. Riguardo alla questione sollevata relativa alle esercitazioni militari che si tengono periodicamente sul territorio sardo, si tratta di attività addestrative indispensabili a conseguire quelle capacità operative che sono requisito imprescindibile di uno strumento militare moderno ed efficace, il cui mandato di difesa della nazione, dei suoi confini e della collettività, discende direttamente dal dettato costituzionale. L'addestramento riveste un'importanza primaria nell'ottica di disporre, a carattere continuativo, di aliquote di forza a differenti livelli di prontezza, in grado di integrarsi rapidamente e di interoperare efficacemente nell'ambito dei dispositivi interforze e multinazionali. Le attività addestrative vengono, comunque, sempre effettuate nel pieno rispetto di precise norme di sicurezza volte ad assicurare la salvaguardia della popolazione, la tutela dell'ambiente e, in generale, di tutti gli operatori durante questa attività. Per quanto concerne, più in particolare, le esercitazioni svolte presso i poligoni, ogni attività è preceduta da un'approfondita analisi dell'impatto ambientale. Inoltre, il reparto utilizzatore della struttura deve: comunicare alla direzione del poligono il tipo di armi e munizioni che prevede di impiegare, prima di ottenere l'autorizzazione e condurre le esercitazioni; presentare, al termine delle attività, un rapporto che conferma l'avvenuta bonifica delle aree utilizzate, il numero e il tipo di munizionamento effettivamente impiegato durante l'esercitazione; adottare parametri da sottoporre di volta in volta ai comandi dei poligoni stessi ai fini della necessaria autorizzazione. Inoltre, al fine di adottare le necessarie misure di sicurezza in mare e di garantire la sicurezza della navigazione, le competenti autorità marittime emanano preventivamente appositi provvedimenti di interdizione degli specchi acque interessati dalle attività di tiro presso i poligoni a mare. Pertanto, il complesso delle misure di carattere preventivo poste alla base delle attività addestrative, e la natura stessa di tali attività, escludono la sussistenza di elementi tali da indurre alla sospensione immediata delle esercitazioni in programma, come auspicato dai senatori interroganti. Ciò detto, non si mette certo in dubbio che lo svolgimento di tali attività possa comportare ripercussioni sul contesto territoriale e sotto diversi aspetti. La Difesa, per compensare tali ripercussioni, opera attraverso vari istituti, organismi e procedure per mitigare l'impatto sulla cittadinanza. In tale ambito, fondamentale è il ruolo dei comitati misti paritetici ove la realtà regionale e le esigenze militari trovano il corretto alveo di confronto e di decisioni concordate in merito alle servitù militari e all'uso dei poligoni. Le attività da svolgere in poligono vengono, infatti, preventivamente valutate e autorizzate solo dopo un esame dell'impatto ambientale e previa consultazione del Comitato misto paritetico costituito presso la Regione Sardegna ai sensi della legge n. 898 del 1976. L'attività di tali comitati è finalizzata proprio ad instaurare nell'ambito di ogni Regione un rapporto permanente di collaborazione con le Forze armate al fine di armonizzare le esigenze della Difesa con quelle del tessuto civile e sociale della vita comunitaria. Continuando la disamina delle questioni sollevate con l'atto in esame, passiamo a trattare il punto relativo all'opportunità di avviare una rimodulazione dello strumento militare non solo in termini di forza e di organizzazione ma anche di compiti in chiave internazionale. Nel merito, sono necessarie alcune considerazioni di carattere generale sull'attuale quadro internazionale e geostrategico, che impone scelte precise in materia di politica di difesa. La tutela della sicurezza nazionale contempla, oltre alla difesa della sovranità nazionale, il concorso alla stabilità e alla sicurezza internazionale, la legittima salvaguardia e la tutela dei nostri interessi nonché la prevenzione dei rischi e il contrasto alle violazioni del diritto e della pace. Tale concetto si fonda sempre più nell'azione delle grandi organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte attiva e responsabile: Nazioni Unite, Unione Europea, Alleanza Atlantica, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nelle quali si incardina, in maniera attiva e responsabile, la sicurezza fondamento della democrazia, del benessere e della coesione nazionale. Il nuovo scenario internazionale impone una continua e attenta rivalutazione della priorità di difesa. Alla luce di tale esigenza, le Forze armate italiane stanno evolvendo dalla dimensione prevalentemente statica della difesa della sovranità verso il sostegno dinamico all'azione della comunità internazionale per la prevenzione e la gestione delle crisi con compiti di pace e sicurezza. La partecipazione dell'Italia alle missioni UNIFIL rappresenta un tangibile esempio di tale evoluzione. Tali impegni devono essere sostenuti con un apparato militare moderno, integrato ed interoperabile con quello dei principali alleati che rendono necessarie scelte coerenti ed efficaci. efficaci. In tale contesto di difesa della pace e di mantenimento della sicurezza, vanno inquadrate le esercitazioni condotte in ambito di *peace* *support* *operations*. Esse assumono notevole rilevanza, in quanto funzionali ad operare nell'ambito delle operazioni discendenti dagli impegni assunti in campo internazionale e nell'ambito delle diverse organizzazioni cui l'Italia aderisce a pieno titolo. Tali esercitazioni apportano un contributo fondamentale nelle operazioni di risposta a situazioni di crisi sotto l'egida dell'ONU a sostegno della stabilità internazionale. A tal fine, si ricerca la massima standardizzazione operativa per migliorare la sicurezza e l'efficacia dei mezzi e la massima capacità di tutti i Paesi partecipanti a questo tipo di attività, che può svolgersi anche con Paesi non necessariamente appartenenti alla NATO. Venendo alla questione della bonifica delle acque e dei fondali marini da ordigni ovvero da materiali esplodenti ad essi assimilabili, la normativa vigente stabilisce che interventi di tale natura siano suddivisi in occasionali e sistematici. In particolare, la bonifica sistematica a scopo preventivo sui fondali marini è effettuata da ditte specializzate, certificate e autorizzate dall'amministrazione militare alla sola fase di ricerca e di localizzazione su mandato della competente autorità territoriale. Non esiste, pertanto, una diretta competenza della Difesa la quale, tuttavia, può intervenire, su formale richiesta, per rimuovere e rendere inoffensivi gli ordigni rinvenuti nel corso delle ricerche sistematiche effettuate dalle ditte autorizzate a tal fine o quelli trovati occasionalmente. Quanto alla bonifica dei fondali e delle acque prospicienti la Sardegna, auspicata dagli interroganti, relativamente al poligono di Capo Teulada sono in corso contatti tra la competente Direzione Generale degli Armamenti Navali ed il ed il *Undersea Research Center* (NURC), al fine di individuare la fattispecie contrattuale attraverso la quale disciplinare le attività di ricerca propedeutiche alla bonifica. Nella zona di Capo San Lorenzo (area del poligono interforze del Salto di Quirra), invece, è stata eseguita in passato una ricerca idraulica tramite intervento di sommozzatori della Marina militare italiana. Va detto, tuttavia, che la quasi totalità dei residui delle attività esercitative svolte dal FISC del Salto di Quirra sono di tipo ferroso ed inerte. Per quanto concerne, ora, la tipologia di addestramento svolto presso il poligono di Capo Frasca, premesso che l'Italia non ha stipulato nessun accordo segreto per il dispiegamento di armi nucleari, denominato Stone Ax, si precisa che i reparti dell'Aeronautica Militare vi si addestrano impiegando esclusivamente armamento da esercitazione di tipo «inerte». Passiamo, quindi, ad analizzare l'aspetto concernente i costi a carico degli utenti per l'utilizzo dei poligoni. Per le aziende produttrici di armamenti, i costi variano sensibilmente in funzione del tipo di risorse impiegate, sia in termini di apparecchiature che di personale; la cifra indicata dai senatori interroganti può essere considerata valida come costo medio orario, in quanto non riferita ad una specifica attività. Le somme direttamente riscosse a seguito delle convenzioni stipulate dalla Difesa con le ditte che utilizzano i poligoni per attività sperimentali sono versate direttamente all'Erario. Le ditte, inoltre, sono tenute a: comunicare al Comando del Poligono il programma delle attività addestrative che, successivamente, viene sottoposto all'approvazione del Co.Mi.Pa (Comitato paritetico Regioni Difesa), a cura delle Autorità militari; redigere, al termine dell'attività, il verbale che attesti l'avvenuta bonifica delle aree utilizzate. Circa, invece, l'aspetto inerente i costi a carico degli Stati stranieri, non è previsto il pagamento di una specifica quota di affitto, ma i costi di utilizzo variano a seconda della tipologia di esercitazione. In particolare, per le esercitazioni NATO, l'aspetto economico è regolato dagli accordi internazionali di standardizzazione. Il rimborso dei costi sostenuti per l'utilizzo dei poligoni differisce di volta in volta. Nel caso in cui la forza armata straniera partecipi ad attività addestrativa congiunta si provvede al recupero dei costi logistici, mentre, qualora venga richiesto l'utilizzo dell'installazione militare per proprie esigenze, si provvede al recupero dei costi logistici e del costo operativo d'impiego del poligono utilizzato, nonché al rimborso di eventuali danni. Di tutte le somme direttamente riscosse si procede al versamento diretto all'Erario. In conclusione, si rassicurano i senatori interroganti riguardo al fermo intendimento della Difesa a voler proseguire, senza alcun pregiudizio e con la massima trasparenza, nell'impegno indirizzato ad armonizzare i molteplici aspetti che attengono alla sicurezza, all'impatto ambientale ed allo sviluppo turistico ed economico delle aree interessate.

ma ho avuto occasione di visitare alcuni di questi poligoni e anche di parlare con le comunità locali a Capo Teulada, a Capo Frasca, al Salto di Quirra. Indubbiamente, da un certo punto di vista, l'impegno a svolgere la seconda conferenza sulle servitù militari è un passo in avanti. Ricordo anche che era un impegno preso dal programma di Governo. Ma d'altra parte, vi sono alcune questioni che a mio parere, motivano la mia insoddisfazione, che riguardano alcuni elementi più concreti

che, in effetti, quelle acque siano piene di residui bellici da esercitazioni, quindi sarebbe utile un confronto a tale riguardo. È anche vero che l'accordo firmato il 10 novembre scorso con il governatore Soru, riguardante alcune aree di demanio militare a Cagliari, è un passo in avanti notevole ed importante; oggi c'è un incontro anche sulla questione dell'arsenale della Maddalena, il 19 dicembre si parlerà anche di Capo Frasca e di Capo Teulada. Ci sono alcune questioni che però, a mio parere, necessitano di una maggiore definizione, ad esempio l'onere relativo alla bonifica, cioè il rispetto del principio internazionalmente riconosciuto del "*polluter pay*", cioè chi inquina paga; in effetti, sarebbe molto opportuno che i costi della bonifica non ricadessero né sulla Regione Sardegna né sulla collettività, che comunque ha già sofferto questa presenza di servitù. Altra questione, a nostro parere importante, è quella di una diversa impostazione,

in Sardegna praticamente c'è la stragrande maggioranza delle servitù militari e del demanio militare rispetto al resto del continente e quindi sarebbe necessario non soltanto parlare di una riallocazione e ridefinizione delle servitù, ma anche di una riduzione di alcune delle spese, secondo un principio che state seguendo e che a mio parere dovrebbe vedere maggiormente coinvolte anche le comunità locali. poi un problema relativo alle informazioni sul munizionamento utilizzato; ho avuto occasione di constatare, anche con della documentazione, che in alcuni casi l'informazione *ex post* è mancata e, comunque sia, mentre è stato ottemperato l'obbligo di fornire la tipologia di munizionamento, dei sistemi d'arma previsti per le esercitazioni, in alcuni casi, invece, questo non è stato accompagnato da un'informativa dettagliata

quella della destinazione di uso finale delle aree liberate, ad esempio sarà molto interessante sapere quale sarà la decisione sull'arsenale della Maddalena; a nostro parere, le aree liberate possono essere restituite alla collettività attraverso un processo che anche il Governo può sostenere, e non soltanto il Ministero della difesa, ma anche i Ministeri per i beni culturali, dell'ambiente e delle attività produttive, per per elaborare delle strategie di riconversione di queste aree che vedano anche la possibilità di riconvertirle in processi produttivi o di generazione di impiego che siano innovativi dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Questo, secondo me, è un elemento sul quale bisogna

che permetta l'uso e la presenza di bombe sul territorio nazionale. A quanto mi risulta, sia a Ghedi che ad Aviano, sono stoccati 90 ordigni nucleari, alcuni gestiti direttamente dagli Stati Uniti, altri, come appunto quelli di Ghedi, che invece possono essere utilizzati, in alcune determinate circostanze, anche dall'Aeronautica militare italiana. Questo è un punto su cui chiederemo un maggiore chiarimento, perché a nostro parere la presenza di quegli ordigni nucleari, mai smentita sino ad rappresenta una grave violazione dell'accordo di non proliferazione nucleare e quindi pregiudica anche il ruolo che l'Italia può e vuole svolgere per il disarmo e la non proliferazione nucleare.

è il soggetto responsabile del Patto territoriale di Ragusa, approvato con decreto del Ministero del bilancio e della programmazione economica in data 27 novembre 2000. Il Patto territoriale di Ragusa, ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, è l'espressione del partenariato sociale per l'attuazione di un programma di interventi nei settori dell'industria, dell'agroindustria ed in quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati, ed è l'accordo tra i soggetti sottoscrittori, ossia enti locali, organizzazioni di categoria, privati beneficiari e non. Il Patto in questione prevede investimenti per euro 79.882.454, con un onere a carico dello Stato di euro di 47.387.502, un capitale proprio investito

Ciò premesso, si fa presente che in merito alla richiesta avanzata dalla SOSVI al Ministero delle attività produttive - così allora si chiamava - in data 12 novembre 2004, concernente l'autorizzazione a rimodulare le risorse derivanti da rinunce, revoche e/o economie conseguite in sede di attuazione del Patto, il predetto Ministero ha verificato la sussistenza dei requisiti di efficienza e di efficacia dell'attuazione del Patto stesso ed ha chiesto alla Regione Siciliana, in data 23 febbraio 2005, il nulla osta a concedere tale autorizzazione. Contrariamente a quanto si afferma nell'atto in esame, la data del 23 febbraio 2005 è, dunque, quella in cui il Ministero ha richiesto il previo parere all'autorizzazione alla Regione Siciliana, non certo quella di un'approvazione che non è mai intervenuta. Riguardo al mancato finanziamento delle rimodulazioni dei Patti territoriali, compreso il Patto territoriale di Ragusa, di cui ci stiamo occupando, occorre precisare quanto La legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero la legge finanziaria 2006, ha previsto una riduzione di 560 milioni di euro delle autorizzazioni di spesa precedentemente disposte per interventi della programmazione negoziata, che si aggiunge a quella di 30 milioni di euro apportata dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35, del 14 marzo 2005, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 80, del 14 maggio 2005.

almeno parziale, del drastico taglio dei fondi operato indistintamente dalla legge finanziaria per il 2006 su tutto il comparto della programmazione negoziata, che ha determinato appunto quel mancato finanziamento. Ai sensi dello stesso articolo 8, le risorse disponibili, in quanto inferiori alle richieste, sono state destinate in via prioritaria alla copertura dei Contratti di programma e non sono residuate risorse per gli altri strumenti della Programmazione negoziata quali i Patti territoriali e i Contratti d'area. Conseguentemente, anche per la rimodulazione del Patto territoriale di Ragusa, che avrebbe dovuto essere finanziata dalle risorse rivenienti da revoche di contributi concessi per iniziative dello stesso Patto, non esistono al momento disponibilità, giacché il taglio di cui si è precedentemente detto è intervenuto in maniera indistinta su tutti gli strumenti della Programmazione negoziata. Per tale motivo, il Ministero non aveva mai formalmente autorizzato la riassegnazione delle risorse alla SOSVI, soggetto responsabile del Patto. Si aggiunge, inoltre, che al 31 dicembre 2006, per disposizione comunitaria, decadranno tutti i regimi di aiuto già autorizzati dalla Commissione europea e quelli da applicare a partire dal prossimo anno dovranno conformarsi ai nuovi orientamenti comunitari validi per il periodo compreso tra il 2007 ed il 2013. L'eventuale finanziamento della rimodulazione del Patto al nostro esame potrà quindi intervenire con le risorse disponibili per il prossimo esercizio finanziario e previa ridefinizione del regime di aiuto secondo la nuova normativa comunitaria.

Governo precedente che, con una disposizione inserita nella legge finanziaria, ha fatto giustizia sommaria di tante positive esperienze a sostegno delle piccole e medie imprese presenti in alcune realtà del Mezzogiorno, tra cui la Provincia di Ragusa.

si è occupata della gestione del Patto territoriale, contava per completare il programma a sostegno di alcune iniziative imprenditoriali. Il relativo *iter* era stato avviato nei tempi giusti si era ottenuta una valutazione positiva da parte del Ministero. Al riguardo, concordo con lei che non si trattava di una autorizzazione, ma di una valutazione positiva, subordinata al nulla osta della Regione siciliana a seguito dell'intervenuta regionalizzazione della

di una pratica fondata su un'efficace azione della società che gestisce il Patto, come lei ha detto,

dicembre, fino a quando, con la legge finanziaria, si è utilizzata questa tagliola. Adesso, signor Sottosegretario, è del tutto evidente che non posso che dichiararmi soddisfatto della risposta e, purtroppo, insoddisfatto dall'esito della vicenda. Confido che il Governo possa attivare tutto quanto è utile affinché, in linea con le nuove regole comunitarie, nel 2007 si possa recuperare questa somma e rendere quindi giustizia ad un territorio che confidava in questi finanziamenti per completare il proprio programma.